la stazione di Rovigo è stata oggetto di lavori di riqualificazione eseguiti da Centostazioni, società del Gruppo Ferrovie dello Stato. Si tratta di interventi che hanno riguardato il fabbricato viaggiatori, con particolare riferimento all'atrio di stazione, e che sono consistiti nel riordino degli spazi interni, nel rifacimento delle pavimentazioni e dei rivestimenti e nella messa a norma degli impianti; sono stati anche completamente ristrutturati i servizi igienici della stazione. Nell'ottica del miglioramento delle condizioni di accessibilità alla stazione e nell'ambito di una prima fase di interventi, sono stati anche realizzati percorsi tattili in continuità con quelli esterni del piazzale. Tutti questi lavori sono stati svolti d'intesa con RFI che, in qualità di proprietaria, ha approvato i progetti ed erogato parte dei finanziamenti necessari. Ora, con i finanziamenti di RFI già stanziati, nel 2017 sarà possibile avviare la seconda fase degli interventi finalizzati a migliorare le condizioni di accessibilità, in particolare i lavori di innalzamento dei marciapiedi di stazione all'altezza *standard* di 55 centimetri di altezza dal piano delle rotaie e, nell'ambito dell'impegno di eliminazione delle barriere architettoniche, anche la realizzazione di ascensori su ciascun marciapiede di stazione. Sulle nuove pavimentazioni dei marciapiedi saranno ovviamente posati i percorsi tattili per ipovedenti,

si tratta, infatti, di lavori complessi che dovranno essere eseguiti compatibilmente con la circolazione ferroviaria e con tempi di esecuzione condizionati dalla necessità di garantire il contemporaneo esercizio ferroviario. Naturalmente, con la realizzazione degli ascensori non sarà più necessario attraversare i binari sulle passatoie a raso per accompagnare ai diversi marciapiedi le persone a ridotta mobilità; va tuttavia puntualizzato che tale operazione - da effettuare finché non saranno disponibili gli ascensori - viene oggi svolta in totale sicurezza mediante l'impiego di personale appositamente abilitato e nel rispetto di precise procedure di sicurezza. Il MIT, dal canto suo, effettuerà ogni necessario approfondimento affinché RFI provveda all'adeguamento della struttura ferroviaria di Rovigo in maniera compiuta.

debbo accogliere con soddisfazione questa risposta, quindi sono anche tenuto a prendere in seria considerazione i tempi che mi sono stati enunciati poc'anzi, per cui li ripeto per rincuorare tutte quelle persone che negli anni hanno subito questo disagio. Le

52 gradini - che ho definito "di indifferenza al problema altrui " - che a molte persone con valige, ma anche a bambini, mamme con carrozzine, anziani, persone normalissime,

contribuito a questo impegno da parte del Governo, che mi auguro venga mantenuto, perché io chiaramente renderò pubblica la promessa

finestra") sull'utilizzo di edifici alternativi alle scuole per le consultazioni elettorali. il senatore Orellana richiama l'attenzione sulle doglianze - riprese anche da alcuni organi di stampa - espresse dall'Associazione nazionale presidi, dal corpo docente e dai genitori per i disagi causati dall'interruzione delle lezioni scolastiche in concomitanza con le consultazioni elettorali e referendarie. Chiede, quindi, che venga accolta la proposta della citata Associazione dei presidi di realizzare un'anagrafe degli edifici pubblici, allo scopo di individuare sedi alternative agli edifici scolastici, idonee all'allestimento dei seggi elettorali, così da non ledere il diritto all'istruzione degli studenti. Il problema evidenziato è noto al Ministero dell'interno che se ne era già occupato, unitamente al Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca, nell'intento quantomeno di ridimensionarne la portata. Più precisamente, i due Dicasteri hanno avviato tempo fa, tramite i Comuni e le prefetture, un'indagine per individuare degli edifici pubblici che potessero sostituire integralmente i plessi scolastici come sedi degli uffici elettorali di sezione in tutto il territorio nazionale. L'iniziativa, tuttavia, con molta franchezza, non ha avuto alcun seguito, essendo emerso un numero assolutamente insufficiente di strutture extrascolastiche idonee allo scopo. Ad oggi, su un totale di 61.553 sezioni su base nazionale, sono 6.979 (cioè 1'11,34 per cento) le sezioni ubicate in edifici extrascolastici.

da parte delle Amministrazioni comunali, di non coinvolgere gli edifici scolastici nell'organizzazione delle consultazioni popolari, ovviamente nei casi in cui ciò risulti materialmente possibile per la presenza di edifici pubblici alternativi. Quanto poi alla scelta del tipo di scuola (dell'infanzia, primaria o secondaria) o comunque dell'edificio sede di seggio, ricordo che (ai sensi del combinato disposto dell'articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 e dell'articolo 26, comma 13, della legge n. 340 del 2000) il luogo di riunione delle sezioni elettorali è stabilito in sede locale dall'ufficiale elettorale di ogni Comune, tenendo ovviamente conto delle esigenze del rispettivo territorio e della condizione dei luoghi.

Signor Presidente, onorevoli senatori, considerata l'analogia delle questioni rappresentate dai senatori interroganti, ho ritenuto opportuno fornire una risposta congiunta. Per prima cosa mi preme evidenziare che, a tutela dell'immagine dei nostri prodotti, della nostra tradizione lattiero-casearia e innanzitutto per una corretta informazione ai consumatori, abbiamo sempre sostenuto, in tutte le sedi nazionali, europee ed internazionali, l'obbligo di indicare in etichetta l'origine dei prodotti e delle materie prime utilizzate per la loro fabbricazione. È ora scattato il via libera europeo allo schema di decreto che introduce l'indicazione obbligatoria dell'origine per i prodotti lattiero-caseari in Italia. La Commissione europea, infatti, non ha sollevato rilievi o obiezioni entro il termine previsto. Questo sistema, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017, consentirà di indicare con chiarezza al consumatore la provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini. Si tratta di un passo atteso da anni, che ci consentirà di valorizzare il lavoro dei nostri allevatori e di tutta la filiera lattiero-casearia. L'Italia si pone all'avanguardia in una sperimentazione sulla massima trasparenza dell'informazione al consumatore. Il nostro obiettivo è che questa norma sia poi estesa a tutta l'Unione europea, dando così più strumenti di competitività e tutela del reddito ai produttori. Il decreto prevede in particolare che il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l'origine della materia prima in etichetta, in particolare indicando sempre il Paese di mungitura del latte. Sono esclusi solo i prodotti DOP e IGP, che hanno già disciplinari relativi anche all'origine, e il latte fresco già tracciato. Per quanto concerne il richiamo alla World Trade Organization (WTO) per proteggere l'identità territoriale degli alimenti, segnalo che tale accordo non regola le problematiche dell'etichettatura dei prodotti. In tale contesto, invero, le valutazioni sulle regole di etichettatura intervengono qualora uno Stato ritenga restrittive per il commercio le norme imposte da un altro membro.

Tuttavia, nella mia interrogazione sollevavo un altro tema e richiamavo espressamente la diffida che la Commissione europea ha inviato all'Italia in merito alla

di polveri di latte per produrre formaggi, yogurt, latte alimentare a tutti i caseifici situati sul nostro territorio nazionale. Rispetto a tale procedura di diffida, Vice Ministro, non ho sentito un resoconto di come stiano andando le cose e non ho avuto una risposta precisa in merito a questa vicenda. Ricordo che la Commissione europea ha ritenuto che la nostra legge nazionale che tutela la qualità delle produzioni, rappresenti una restrizione della libera circolazione delle merci, essendo invece la polvere di latte e il latte concentrato utilizzati in tutta Europa. A nostro avviso questo è molto pericoloso ed io sottolineavo una presa di posizione forte di tutte le associazioni di categoria, in particolare del settore lattiero caseario, proprio a significare la forte preoccupazione, che in me permane e credo permanga in tutto il settore, finché non vi sarà

Sono consapevole che questa normativa non intacca l'economia dei formaggi DOP perché, come lei ricordava, vi sono disciplinari di produzione già ben chiari che fanno riferimento a origine e qualità del latte. Tuttavia, rimane una forte preoccupazione per tutte le altre produzioni, che rappresentano il 50 per cento - lo voglio ricordare - del prodotto lattiero-caseario italiano. Questa normativa, cioè l'imposizione da parte dell'Europa all'Italia di togliere questo divieto e quindi di entrare in un meccanismo di produzione allargata, per cui questi prodotti in polvere e derivati vengono messi in commercio, potrebbe assestare quello che io chiamo un colpo decisivo che può mettere a repentaglio il lavoro dei nostri allevatori. Fra l'altro, ricordo che i produttori di latte - come lei immagino saprà bene - sono già in forte sofferenza economica anche a causa del prezzo del latte alla stalla, che viene pagato, diversamente da altri Paesi, soprattutto del Nord Europa, in maniera molto discriminatoria: in Veneto dai 32 ai 38 centesimi per litro, che non è nemmeno sufficiente a coprire i costi di produzione. Registriamo un continuo chiudersi di stalle, con tutti i problemi connessi, perché poi ne deriva un grave danno per tutto l'indotto.

europea - azioni urgenti e precise che vadano a contrastare questa costituzione in mora e che possano difendere davvero le produzioni e la qualità dei nostri prodotti. Ricordo l'eccellenza del nostro *made in Italy* e dei nostri prodotti

la disponibilità del Governo a tutelare l'immagine del prodotto italiano, con l'obbligo dell'indicazione di origine del latte e della materia prima, che è un fatto molto importante, richiesto fortemente da tutte le associazione di categoria.

e i produttori di prodotti caseari sono migliaia. Vengo da una Regione, la Puglia, che produce in notevole quantità prodotti produttori, dunque, non possono che cercare di avere dal Governo un sostegno nella difesa della loro specificità e della loro qualità,

Signor Presidente, onorevoli senatori, la normativa nazionale concernente la materia in parola è allineata al quadro normativo sovranazionale, in particolare al dispositivo degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 1627 del regolamento n. 1627 del 2016. I provvedimenti nazionali sulla ripartizione del contingente di cattura del tonno rosso,

Il regolamento n. 1627 del 2016 ha recepito le disposizioni della raccomandazione ICCAT 14-04, vincolante per l'Unione europea. Tale norma sovranazionale, pur prevedendo l'incremento progressivo del Total Allowable Catch (TAC) ha inteso comunque mantenere un approccio precauzionale nella gestione del rapporto tra possibilità e capacità di pesca. Ciò al fine di evitare che i benefici (in termini di conservazione e ricostituzione degli *stock*) derivanti dai più stringenti piani pluriennali applicati nel precedente quinquennio 2010-2014 potessero essere inficiati da un numero troppo elevato di operatori autorizzati. Benché tale limite numerico (peraltro, ancor più stringente per il settore specifico della "circuizione"), in via del tutto eccezionale e/o residuale, può essere derogato qualora la parte contraente e/o lo Stato membro dimostri l'impossibilità di poter sfruttare integralmente il contingente di cattura assegnato, rilevo che tale circostanza non si è mai verificata per le flotte nazionali annualmente autorizzate alla cattura bersaglio del tonno rosso. Le legittime aspettative delle marinerie non espressamente autorizzate alla cattura bersaglio del tonno rosso (ivi comprese quelle artigianali), vengono soddisfatte attraverso le catture accessorie. Al riguardo evidenzio, per la prossima campagna di pesca, l'ulteriore incremento, rispetto al 2016, del relativo *plafond* nonché la possibile conferma (ove ne ricorrano i presupposti) di un ampliamento del limite annuale, come già operato nel corso del 2016 con il decreto ministeriale 5 aprile 2016,

Signor Vice Ministro, grazie per la sua pronta risposta alla nostra interrogazione. Mi spiace, però, dover confermare che non mi ritengo pienamente soddisfatta dalla scelta, adottata anche quest'anno, di confermare solo i quarantadue pescherecci già autorizzati per la pesca al tonno rosso,

Confermando, infatti, questa scelta, si tutela e rispetta la dinamica dello *stock* ittico. Quindi, si rispettano pienamente le prescrizioni del regolamento dell'Unione europea n. 1627 del 2016, ma si continua a trascurare il sostegno alle imprese di piccola pesca artigianale, sostegno previsto all'articolo 8 del regolamento citato precedentemente. Aggiungo, inoltre, che nel decreto del MIPAAF del 17 maggio 2015, al paragrafo 3 dell'articolo 2, si prevede espressamente che se il quadro se il quadro tecnico-giuridico fosse cambiato in seguito a mutamenti di normativa (avvenuti proprio con il regolamento UE 1627 ) si sarebbe provveduto a modificare le tabelle di ripartizione fra i singoli sistemi. purtroppo, constato che ciò non è avvenuto; soprattutto se poi si considera che nell'attuare il piano di ricostituzione, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere attività di pesca costiera e l'utilizzo di attrezzi e tecniche di pesca selettivi, caratterizzati da un ridotto impatto ambientale, compresi gli attrezzi e le tecniche utilizzati nella pesca artigianale e tradizionale, e soprattutto indirizzando gli Stati membri a limitare l'aumento delle quote alla circuizione, indicata come il sistema più distruttivo della pesca del tonno. Visto che la circuizione li cattura proprio nel periodo della riproduzione, non si capisce perché non si possano ripartire gli aumenti alle imbarcazioni della pesca artigianale per "contribuire ad un equo tenore di vita per le economie locali". Come abbiamo sostenuto più volte nel corso del nostro mandato, sia la sottoscritta che gli altri firmatari della interrogazione, le quote delle catture accessorie effettuate dalle imprese liguri e sarde nello specifico, vengono giudicate insufficienti per il prosieguo dell'attività economica da parte degli operatori, operatori che il regolamento UE vorrebbe tutelare. In conclusione, si invita nuovamente a riconsiderare i regimi di autorizzazione adottati al fine di poter distribuire gli eventuali aumenti futuri di quote

Infatti, a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, si è delineata in modo chiaro e inequivocabile

i poteri di vigilanza e controllo sulle modalità organizzative e di funzionamento delle aziende sanitarie e alle aziende stesse, nella figura del direttore generale, la responsabilità gestionale e organizzativa. Pertanto, la gestione delle procedure concorsuali e delle relative assunzioni rientra nella specifica attività, competenza e responsabilità dell'azienda sanitaria di riferimento che, in quanto tale, ha il dovere di effettuare gli opportuni controlli rispetto alla veridicità

Fatta questa doverosa precisazione e passando nello specifico al caso che qui interessa, fornisco, di seguito, gli elementi pervenuti, per il tramite della competente prefettura, dall'assessorato alla salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento. In primo luogo, si fa presente che l'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento ha segnalato il presunto mancato conseguimento della laurea e dell'abilitazione professionale del signor A. S. ai competenti organi giudiziari, fornendo agli stessi i documenti richiesti per lo svolgimento delle attività in corso. Inoltre, l'azienda ha provveduto a comunicare alla procura della Corte dei conti gli elementi utili per la valutazione del danno sofferto dall'azienda provinciale, qualora i fatti addebitati alla persona in questione risultassero accertati.

deliberazione n. 1423 del 2004 in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, in occasione di nuove assunzioni l'amministrazione pone in essere una verifica sistematica, con controlli cosiddetti a tappeto, delle dichiarazioni sostitutive rese. In tali circostanze è prevista la verifica dell'iscrizione all'albo relativamente alle professioni per cui è richiesta l'appartenenza a un ordine professionale e la verifica del possesso del titolo di studio nelle ipotesi in cui quest'ultimo sia diverso da quello necessario per l'iscrizione all'albo (come accade, per esempio, per le specializzazioni), ovvero nelle ipotesi in cui l'assunzione riguardi qualifiche per le quali non è richiesta l'appartenenza a un albo professionale.

all'articolo 2 («Dichiarazioni sostitutive di certificazioni») si prevedeva che fatti, stati e qualità personali, tra i quali le iscrizioni in albi, erano comprovati con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Di qui, il ruolo dell'ordine professionale di riferimento quale garante, da un lato, del corretto esercizio della professione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e, dall'altro, del necessario controllo sui propri iscritti. Per quanto riguarda l'attività prestata in Veneto, si precisa che la medesima Regione, per il tramite della prefettura di Venezia, ha comunicato al Ministero della salute che, con nota del 7 ottobre 2010, «sono state 2010, «sono state impartite alle aziende ed enti del sistema sanitario regionale indicazioni per l'effettuazione delle verifiche, nei confronti del personale dipendente, dei documenti identificativi e dei titoli abilitanti allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo di inquadramento». Inoltre, con riferimento al caso di specie, il direttore generale dell'azienda ULSS di Mirano ha rappresentato che l'attività svolta dal signor A. S. non è stata resa nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, ma rientrava in un piccolo appalto di servizi affidato ad una ditta per l'effettuazione di alcuni turni di guardia medica presso i reparti di pediatria, qualora, in via del tutto eccezionale, a cause delle improvvise carenze di organico risultasse difficoltoso garantire i servizi di guardia. Viene precisato ulteriormente dal medesimo direttore che il capitolato speciale prevede due livelli di controlli in tema di titoli abilitanti del personale: un controllo affidato alla diretta responsabilità dell'appaltatrice ed un controllo svolto dall'azienda ULSS. Quest'ultimo è stato effettuato, nel rispetto di quanto previsto dalle direttive regionali, mediante consultazione diretta dell'Ordine dei medici di Ferrara. Ad ogni modo, stando a quanto riportato dal direttore generale, «il signor A. S. presentava una pluriennale attività di servizio presso enti pubblici ed aziende sanitarie, era ampiamente conosciuto dal personale medico dell'azienda come un professionista esperto nonché dotato di abilitazione primariale (...)». Infine, il direttore generale dell'azienda sanitaria di Bassano del Grappa ha comunicato che «la specializzazione non era richiesta ai fini dell'assunzione sino al 1° febbraio 1998, data in cui è divenuta obbligatoria ai sensi dell'articolo 24 del decreto del con esclusione del personale in servizio di ruolo alla data suddetta. Pertanto, i titoli di cui il signor A. S. doveva obbligatoriamente risultare in possesso ai fini dell'assunzione si limitavano alla laurea, all'abilitazione all'esercizio della professione e all'iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, la quale a sua volta sottende il possesso dei precedenti due titoli quali requisiti imprescindibili». Da ultimo, ma non per questo meno importante, ritengo doveroso segnalare che il medesimo direttore dell'ASL ha comunicato che il signor A. S. non ha mai ricoperto ruoli di responsabilità apicale presso l'azienda e comunque di essere in possesso non solo di copie conformi dei certificati di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione, autenticate da un notaio, «ma anche e soprattutto del certificato in originale rilasciato dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Ferrara», dal quale risulta la data di conseguimento della laurea, dell'abilitazione all'esercizio della professione e dell'iscrizione all'albo professionale. Il caso è aperto.

Nel merito, voglio rileggermi la risposta per capire bene, perché alcuni passaggi lasciano ancora il mistero intorno a questa situazione verificatasi in Trentino e in Veneto. Peraltro c'è un procedimento mi risulta che nei prossimi giorni ci sarà un dibattimento specifico, quindi lasciamo alla giustizia il compito di fare chiarezza su tutta la vicenda.

quindi è chiaro che c'è una responsabilità personale e una responsabilità delle istituzioni, sia a livello locale, sia a livello nazionale, sulle quali forse da parte nostra è opportuno comunque

si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, sulla base degli elementi pervenuti dalla prefettura di Forlì-Cesena. Come ritenuto dal direttore generale dell'azienda sanitaria locale della Romagna, sul caso specifico richiamato dall'interrogazione, tutti gli operatori - secondo il direttore generale - hanno operato in modo corretto nel rispetto delle linee condivise e consolidate. Lo stesso ha precisato che già dall'anno 2006 in applicazione del progetto regionale PRIMA RER (Progetto infarto miocardico acuto Regione Emilia-Romagna) nel territorio Romagnolo sono state individuate dalla programmazione sanitaria, secondo il modello della rete integrata *hub & spoke*, tre sedi per effettuare gli interventi di angioplastica primaria in corso di IMA Stemi, che sono Forlì, Rimini e Ravenna. Pertanto, l'invio in sala di emodinamica dei pazienti con IMA Stemi dal territorio cesenate segue i criteri di vicinanza, secondo un modello a rete attivo dal 2006, che assegna i casi all'ospedale più vicino tra le sedi *hub* di Rimini o Forlì. Nel corso dei successivi dieci anni, la rete si è ulteriormente sviluppata e sono stati migliorati i percorsi di centralizzazione nelle sedi sopra citate e la competenza dei professionisti che operano in Romagna nel settore dell'emodinamica interventistica, ottenendo risultati molto validi sia in termini di riduzione della mortalità (che non mostra differenze fra i cittadini di Forlì e quelli di Cesena), sia di casi trattati, che di tempi d'intervento quando attivato il 118 nella relazione di emergenza territoriale. L'attività di emodinamica della sede di Forlì vede la partecipazione, già da tempo, dei cardiologi dell'*equipe* di Cesena nell'organizzazione delle attività e delle reperibilità, consentendo una distribuzione delle competenze sul territorio e il mantenimento presso la sede ospedaliera di Cesena dell'offerta di prestazioni programmate di coronarografia e angioplastica entro tempi di attesa congrui, nonché lo sviluppo dell'attività di elettrofisiologia. Questa stretta integrazione, che rappresenta un esempio di sinergia fra *équipe* omogenee, può essere ulteriormente incrementato e costituisce un modello organizzativo valido anche per le altre branche specialistiche, in un'ottica di corretto equilibrio fra efficacia ed efficienza da una parte e sostenibilità dall'altra. Gli indicatori che sono stati richiamati dalla Commissione cardiologica e cardiochirurgica regionale nel documento del settembre 2014, dalla delibera regionale 2040 del dicembre 2015, contenente le linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete ospedaliera secondo gli *standard* previsti dalla legge n. 135 del 2012, dal patto per la salute 2014-2016 e dal 2015, confermano la validità del modello attuale della Romagna, che è stato oggetto di presentazione e dibattito più volte in occasione di confronti pubblici, fra cui la quarta commissione consigliare del Comune di Cesena, il 20 maggio 2015 e la conferenza stampa dell'8 agosto 2016. Nello specifico, per l'ambito di Cesena-Forlì, all'interno del modello della rete assistenziale cardiologica, le linee di sviluppo messe in campo per il 2016 dal dipartimento cardiovascolare dell'ASL della Romagna riguardano il potenziamento dell'attività programmata presso Cesena e ulteriori sinergie che si potranno realizzare con l'integrazione delle competenze professionali e dell'offerta con l'*équipe* della sede all'interno di un progetto complessivo che ha l'obiettivo di rendere equo l'accesso alla cure a tutti i cittadini, indipendentemente dall'area geografica di residenza. Ringrazio il Ministero della salute, qui rappresentato dal sottosegretario De Filippo, per l'attenzione che ha voluto dedicare al caso relativo al decesso di un paziente durante il trasporto tra l'ospedale Bufalini di Cesena e l'Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. Ciò detto, posso ritenermi solo parzialmente soddisfatta dalla risposta ricevuta in quanto il problema della riduzione sconsiderata di stanziamenti a cui è soggetta la sanità pubblica, che non ha trovato lo spazio adeguato nella risposta del Sottosegretario, ha creato, crea e creerà ancora molte tragiche situazioni, quale quella appena ricordata: di questo dobbiamo essere tutti ben consapevoli. La cattiva interpretazione della *spending review* in ambito sanitario sta generando ovunque, nel nostro Paese, situazioni di gravi e gravissimi disservizi, di cui i cittadini sono le vittime predestinate. Pensare che fare *spending review* voglia dire ridurre o quantomeno ridimensionare l'erogazione di salute, piuttosto che affrontare concretamente e sistematicamente la lotta ai numerosi sprechi cui assistiamo giornalmente in ogni ospedale in ogni ASL, è l'unica vera azione che il Ministero dovrebbe attivare. Chiudere una unità di terapia intensiva coronarica, in questo o quell'ospedale, non vuol mai dire risparmiare; comunque - e questo va detto molto chiaramente - i risparmi non si possono mai fare giocando con la vita e la morte delle persone. Quali risparmi effettivi si sono ottenuti? Qualcuno lo ha mai calcolato, sia in termini strettamente economici, sia dal punto di vista del diritto alla salute dei cittadini? Quanto vale una vita perduta? Chi ha deciso di privilegiare la permanenza o l'eliminazione di un servizio in un ospedale e lasciarlo in un altro si è posto solo il problema economico oppure ha studiato le diverse alternative, in modo da poter sempre salvaguardare il bene massimo che è la vita del paziente? Se dovessi dare una risposta, basandomi sul caso di cui stiamo discutendo oggi, dovrei affermare che, evidentemente, ciò non è avvenuto. Voglio ricordare a tutti in quest'Assemblea che la perdita di ogni vita umana andrebbe sempre analizzata a fondo, al fine di evitare il ripetersi, in futuro, di fatti tragici e fatali come quello di Cesena.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con riferimento alle questioni poste dal senatore interrogante, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente con nota del 7 novembre 2016, si rappresenta quanto segue. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha aderito in passato alla fondazione Clinton Global Initiative (citata dall'interrogante come Bill Hillary & Chelsea Clinton Foundation) negli anni 2009-2010-2011-2013, corrispondendo, per ciascuno di questi anni, la quota associativa prevista di 20.000 dollari (ovvero 14.065 euro nel 2009, 14.570,88 euro nel 2010, 14.490 euro nel 2011 e 14.765,59 euro nel 2013). La suddetta organizzazione, fondata dal presidente Clinton quale momento di incontro e scambio tra i Governi, il settore privato e le organizzazioni non governative, investe quattro aree tematiche quali la *economic empowerment*, istruzione, ambiente ed energia e *global dando vita ad azioni di avvicinamento a modelli di sostenibilità ambientale e alla presentazione di progetti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nei Paesi in via di sviluppo, a cui era destinata la contribuzione dell'Italia. I relativi provvedimenti di spesa, emanati con decreto direttoriale negli anni passati, sono stati effettuati a valere sui capitoli di bilancio: 2.214 per gli anni 2009 e 2010, 2.038 per il 2011 e 2.215 per il 2013. Da quanto sopra esposto, si evince, pertanto, che la contribuzione da parte del Ministero è stata interrotta a partire dal 2014, anno di insediamento del presente Governo.

per evitare di entrare, sia pure indirettamente, in un ambito politico di un altro Paese. È infatti ben chiaro che la candidatura di Hillary Clinton non nasce improvvisamente, l'altro ieri, ma è nata molti anni fa, tanto che già nel 2008

Signor Presidente, con riferimento alle questioni connesse alla società Eco Transider Srl di Gricignano di Aversa (Caserta), sulla base degli elementi acquisiti dall'apposita direzione generale del Ministero dell'ambiente e dagli enti territoriali competenti, si rappresenta al senatore Romano e all'Assemblea quanto segue. Occorre, in via preliminare, evidenziare che la competenza in materia di autorizzazione di impianti di gestione dei rifiuti è in carico alle amministrazioni regionali per quanto riguarda, come nel caso di specie, l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. È utile evidenziare inoltre che, ai sensi della normativa ambientale, la competenza territoriale in ordine al controllo delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso anche l'accertamento delle violazioni di cui alla parte quarta del testo unico ambientale, spetta alle Province o alle Regioni alle quali tali poteri potrebbero essere stati ritrasferiti a seguito della loro abolizione. Tali autorità competenti sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti che smaltiscono rifiuti e, ai fini dell'esercizio di tali funzioni, possono anche avvalersi di organismi pubblici, ivi incluse le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente con specifiche esperienze e competenze in materia. Per quanto concerne il caso di specie, si segnala che la ditta è autorizzata in procedura ordinaria regionale, ai sensi dell'articolo 208 del testo unico ambientale, alla gestione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non, nonché alle emissioni in atmosfera e che, in data 5 settembre 2014, la stessa ha presentato istanza volta ad ottenere l'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la quale sono ancora in corso le procedure di autorizzazione. Si rappresenta, inoltre, che, secondo quanto riferito dalla prefettura di Caserta, la società Eco Transider Srl è attualmente sottoposta ad amministrazione controllata, a seguito di un provvedimento di sequestro adottato, in data 10 luglio 2012, dal tribunale di Napoli, e del sequestro preventivo disposto dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 23 settembre 2013. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, l'impianto in questione è stato sottoposto, negli ultimi anni, a numerose attività ispettive da parte dell'ARPA Campania. Nello specifico, secondo quanto riferito dalla predetta agenzia, durante il sopralluogo eseguito in data 29 agosto 2016 dai tecnici dell'ARPAC di Caserta, unitamente al comando di polizia locale di Gricignano di Aversa, sono state riscontrate diverse criticità gestionali connesse allo svolgimento di operazioni non autorizzate, tra cui l'inosservanza delle prescrizioni inerenti i rifiuti pericolosi e non, l'assenza di autorizzazione integrata ambientale e, contemporaneamente, sono state impartite dal personale ARPAC precise prescrizioni per la risoluzione delle criticità riscontrate. È stato prescritto, in particolare, di ripristinare le aree di stoccaggio esterne ed interne all'impianto; di adottare le modalità di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi nel rispetto delle capacità delle singole aree di stoccaggio; di contenere l'altezza dei cumuli come autorizzato; di attenersi al limite quantitativo dei rifiuti stoccabili. Inoltre, per permettere l'effettuazione di un controllo più efficace sul funzionamento dei sistemi di trattamento delle emissioni, l'agenzia ha richiesto alla ditta di implementare l'impianto *scrubber* con un misuratore di portata in continuo in ingresso, con indicatore del numero di ore di funzionamento. Si rappresenta altresì che, al fine di migliorare la qualità delle emissioni, soprattutto quelle con elevato potere osmogeno, il dipartimento dell'ARPAC di Caserta, nelle conferenze di servizi tenutesi per il rilascio degli atti autorizzativi, ha imposto alla ditta la realizzazione di sistemi di abbattimento che, se gestiti adeguatamente, portano ad un netto miglioramento della problematica delle molestie olfattive. Anche la Regione Campania è intervenuta nella vicenda in esame, sia con decreto dirigenziale del novembre 2015 della giunta dipartimento della salute e delle risorse naturali, direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema, con cui ha impartito alla ditta una serie di prescrizioni, sia con atti di diffida emessi successivamente al sequestro giudiziario dell'impianto, nonché in conseguenza dei numerosi sopralluoghi dell'autorità giudiziaria e di controllo. A seguito della comunicazione dell'ARPAC di Caserta degli esiti dell'ultimo sopralluogo effettuato presso l'impianto nel mese di agosto 2016, è in corso di emanazione da parte della competente unità operativa dirigenziale di Caserta della Regione Campania un nuovo atto di diffida che, nelle more della definizione del procedimento penale, ripropone le prescrizioni già impartite, richiedendo nel contempo all'ARPAC l'effettuazione di un nuovo sopralluogo per la verifica di ottemperanza delle stesse.

per complessivi 31.195 metri quadri disposta a favore del consorzio Steel Woman srl e delle sue consorziate, tra le quali figura anche la ditta Eco Transider Srl. Inoltre, al fine di acquisire gli elementi di dettaglio necessari per svolgere le opportune valutazioni in relazione ai possibili profili di danno ambientale,

a trasmettere urgentemente informazioni aggiornate in merito all'attuale stato dei luoghi e alle iniziative intraprese a tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Le informazioni e la documentazione raccolta in riscontro saranno trasmesse all'ISPRA che, su apposito incarico del Ministero, procederà ad elaborare la relazione di valutazione del danno ambientale. Con la medesima nota è stato chiesto all'ARPAC e agli enti locali di continuare a tenere aggiornata la direzione generale del Ministero in merito all'efficacia delle attività di messa in sicurezza e ripristino, individuate nella relazione di sopralluogo dell'ARPAC, cui la ditta deve provvedere a seguito dell'incendio del 5 ottobre ultimo scorso. Infine, con la predetta nota è stato chiesto alla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere di informare il Ministero qualora siano in corso procedimenti penali in merito alla vicenda in argomento. Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, il Ministero continuerà a tenersi informato e continuerà a svolgere un'attività di sollecito nei confronti dei soggetti territorialmente competenti, anche al fine di valutare eventuali coinvolgimenti di altri soggetti istituzionali.

in merito a una vicenda che ha fortemente turbato il territorio non solo del Comune in oggetto, Gricignano di Aversa, ma tutto il circondario. Essa inerisce a un tema molto dibattuto, controverso, direi anche polemico, che riguarda anche il conflitto di competenze che viene a determinarsi su vari territori, nello specifico quello campano, per quanto concerne le responsabilità conseguenti in ambiti che sono di per sé concorrenti. evidente che la salute dei cittadini e la salubrità dell'ambiente sono diritti fondamentali costituzionalmente tutelati, di primaria importanza. E risulta anche evidente come su questo inquinamento atmosferico, definito genericamente come «miasmi»,

questo inquinamento dell'aria non è semplicemente addebitabile a un cattivo odore che proveniva da determinate aziende, ma deve farci interrogare sulle ripercussioni che si possono avere a livello salutare.

rispetto alla quale si evidenzia anche un'assoluta necessità, quella di monitorare continuamente un territorio che già di per sé si è caratterizzato per una storia, nemmeno tanto lontana, di forti inquinamenti estremamente lesivi non solo per la vivibilità, ma anche per la sopravvivenza dei cittadini. Basti dire, senza che questo voglia significare una correlazione diretta tra l'inquinamento di cui abbiamo parlato e i risultati, l'ultimo *report* del registro tumori dell'ASL di Caserta, i cui dati si riferiscono agli anni 2008-2010 (ma sono in corso di aggiornamento per gli anni successivi), per i 104 Comuni della provincia di Caserta - cito in maniera puntuale il *report* stesso - i tassi di incidenza standardizzati di tumori risultano significativamente superiori rispetto al Sud; così per quanto riguarda i tassi di mortalità, sebbene per le donne i tassi risultino inferiori rispetto al Nord. Credo che questo stia ad indicare l'assoluta necessità che la responsabilità,

sia un impegno significativo che mi soddisfa, signor Vice Ministro, per un motivo molto semplice: perché altrimenti i nostri territori continueranno ad essere vessati da episodi gravemente lesivi per l'ambiente